continuare a confondere la realta con la sua rappresentazione. La rappresentazione equella delle dichiarazioni del ministro Tremonti che, a meta settembre, al Meeting di Rimini, affermoche il Governo aveva deciso

sulla defiscalizzazione, sull’aumento degli assegni familiari e delle pensioni, ossia sull’aumento dei redditi di quelle categorie a cui appartengono le famiglie in difficoltain questa situazione di crisi. Vi abbiamo offerto un ventaglio di alternative possibili; nessuna di esse e sta accolta. Pertanto, e` inutile raccomandarsi al Governo.

condivisibile ed efficace, vale a dire la possibilitaper le autonomie locali di rinegoziare i mutui con la Cassa depositi e prestiti, con zero oneri per la finanza pubblica. In un momento di difficolta per gli enti

Da allora, Presidente, sono stati emanati quattro decreti-legge, e rimasta una non sostanziale, ma totale differenza di gestione del regime di restituzione delle imposte per i terremotati abruzzesi rispetto

sia per quanto riguarda i contributi in ambito agricolo, sia per le provvidenze concernenti un evento calamitoso in una Provincia del Veneto.

l’accoglimento come raccomandazione, e una proposta assolutamente surreale, che denuncia in modo molto chiaro la scarsissima considerazione che vi eper le nostre proposte da parte della maggioranza. Non voglio entrare in polemica con nessuno,

Anche in quest’ordine del giorno c’eun impegno di spesa: mi pare quindi che ci sia un doppio peso e una doppia misura nella valutazione. Inoltre, valutazione. Inoltre, voglio dichiarare che, come non ho votato gli emendamenti presentati dal Partito Democratico e dall’UDC, cosı non sono affatto d’accordo su quest’ordine del giorno, per il quale cosıgraziosamente il Governo da la sua disponibilitaad allargare le maglie della spesa, non fosse altro perche´ in questo dibattito non abbiamo ancora ben capito quanto conti la pressione esterna di un certo tipo sul Governo e quanto conti invece l’interesse

sta facendo acqua da tutte le parti e che ha messo la nostra scuola ai margini della scuola europea: e voi vi preoccupate di finanziare le scuole private.

trasformazione in ordine del giorno?

facolta`. LONGO (PdL). Signor Presidente, con il consenso del primo firmatario, senatore Possa, chiedo di poter aggiungere la mia firma all’emendamento 2.381 (testo

quindi sicuramente utilizzabili nel 2010 per far fronte alle esigenze di sviluppo del sistema della ricerca italiana.

di chiedere, nella quota prevista, una parte di questa.

del totale monopolio concesso improvvidamente alle banche per l’asseverazione dei progetti di finanza di progetto. Improvvisamente sono stati esclusi da questa possibilitaaltre categorie, in particolare quella dei revisori dei conti. propone di rimuovere questo monopolio e quanto meno di aprire anche ad altri operatori, come nel caso dei revisori dei conti, la possibilita di asseverare progetti di finanza di progetto. Quindi, non comporta alcun onere ed ein linea con le posizioni del Popolo della Liberta e del Governo in tema di concorrenza e mercato.

ma chiedo al relatore e al Governo un’ulteriore riflessione sull’argomento, e se non valga la pena di sanare subito questo vulnus un po’ strano

Signor Presidente, si tratta di un problema serio che – ahime`! – non si riesce a risolvere in questa sede per gli effetti collaterali che potrebbe produrre. Il Governo si rende conto dell’importanza della questione, ma crede che un ordine del giorno potrebbe aiutare a risolverla. Presidente, l’emendamento 2.432 proponeva l’adeguamento della dotazione di personale dell’Autoritaper l’energia,

A questo punto, francamente sono in imbarazzo, ma per disciplina di Gruppo ed essendo ovviamente convinto sostenitore del Governo,

lo accolga come ordine del giorno.

Di questi ordini del giorno, caro relatore, ne ho presentati una decina. E[ ]inutile ripetere sempre le stesse cose. Credo che sia un problema importante, e non solo

a gente che sta nei cottage, come li chiamate voi, nelle periferie di piccoli paesi di 1.000 abitanti? Si tratta di un cratere di 20.000 abitanti, eppure voi,

nell’istruttoria delle pratiche, cosa che non fate. Bisogna essere severi, condannare e perseguire chi dalle calamitanaturali puo ricavare vantaggi di ordine politico

sono state chieste da ogni parte politica. Vi avevamo invitato a fare delle ispezioni: voi del Governo potete mandare benissimo degli ispettori amministrativi a verificare lo stato della

pochi minuti per spiegare di cosa stiamo parlando, poiche´ a volte certi dinieghi sono veramente incomprensibili e fuori luogo.

Tali Comuni godono, allo stato, esclusivamente del contributo per la ricostruzione privata della prima casa. Gli enti pubblici, invece, non usufruiscono di alcun beneficio tra quelli contenuti nel decreto per il terremoto, per esempio per quel che riguarda gli edifici scolastici, gli edifici pubblici, le infrastrutture pubbliche e cosıvia. Questo emendamento tende a stabilire una cosa semplicissima: per quei Comuni che hanno subıto danni dal terremoto ed esclusivamente per quei danni e solo per il 2010 si deroga dal Patto di stabilita`, con copertura finanziaria prevista sul Fondo contenuto nel decreto n. Francamente non comprendo come la maggioranza e il Governo possano rifiutare una norma come questa, che non puoche produrre

avranno la possibilita di fare con le proprie risorse la riparazione, la messa in sicurezza delle scuole piuttosto che degli edifici pubblici, non graveranno sui fondi per la ricostruzione. Francamente continuo a non comprendere un rifiuto totalmente immotivato, probabilmente dettato dal fatto che non si vuole comprendere qual ela realta di questi Comuni.